Comunico che in data 10 luglio 2018 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri dell'interno; degli affari esteri e della cooperazione internazionale; delle infrastrutture e dei trasporti; e dell'economia e delle finanze* «Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici»

intende perseguire attraverso la crescita delle nostre esportazioni in campo agricolo e alimentare, facendo leva sull'eccellenza delle nostre produzioni, come il vino, di cui siamo primo produttore mondiale. Preso atto dell'interpretazione restrittiva della Commissione europea riguardo a talune disposizioni dei regolamenti n. 1149 del 2016 e n. 1150 del 2016 (che, di fatto, impedivano la prosecuzione delle azioni promozionali nei Paesi terzi ai produttori vinicoli europei che avessero svolto tale attività negli ultimi cinque anni, indipendentemente dal periodo di programmazione), questo Ministero si è attivato, coinvolgendo le delegazioni di Francia e Spagna, per rappresentare le conseguenti ripercussioni negative sul comparto, evidenziando al contempo che, essendo le nuove norme entrate in vigore nel corso del 2016, tale interpretazione avrebbe dovuto acquisire efficacia solo a partire dalla medesima data, consentendo quindi

La Commissione ha inoltre ribadito che l'articolo 4 del citato regolamento delegato n. 1149 del 2016 non dispone l'esclusione l'esclusione dalla misura di sostegno alla promozione prevista dall'OCM Vino per i soggetti beneficiari che abbiano realizzato nei cinque anni operazioni di promozione. La norma vieta ai soggetti ai soggetti proponenti di realizzare una specifica operazione in un determinato mercato di un Paese terzo per un periodo superiore ai cinque anni. La Commissione ha inoltre evidenziato che, superati i cinque anni di operatività in un determinato mercato, al medesimo soggetto è consentito presentare domande di contributo per attività da realizzare in diversi mercati del medesimo Paese terzo o di altri Paesi terzi, oppure realizzare operazioni di tipo diverso nel medesimo mercato del Paese terzo per ulteriori cinque anni. Alla luce anche della precisazione da parte della Commissione che il limite di cinque anni per lo svolgimento di specifiche operazioni di promozione in determinati mercati dei Paesi terzi deve essere comunque verificato dai Paesi membri a partire dalla data di di entrata in vigore del citato regolamento delegato n. 1149, ossia dal 18 luglio 2016, appare chiaro che i soggetti beneficiari che abbiano già in passato realizzato attività di promozione in Paesi terzi, possono continuare a realizzare le medesime operazioni in tali mercati per cinque annualità successive a tale data.

Questa disposizione che la direzione generale per l'agricoltura della Commissione europea ha posto, attraverso una limitazione dello spazio temporale entro il quale è possibile esercitare un'azione di promozione sui mercati esteri, sui mercati esteri, limita fortemente la possibilità di successo dell'azione sui suddetti mercati. Se parliamo di mercati come quello cinese, immaginare che un'azione di promozione possa risolvere la capacità di rendersi attrattivi su quel mercato con una limitazione temporale limitata a cinque anni, secondo me è un errore.

di non immaginare che tale questione sia risolta, perché non lo è affatto. Anzi, semmai, l'intesa che coinvolge la Spagna, che è stata proprio il Paese che ha tentato di utilizzare quella disposizione ministeriale in questo senso, è letale per le attività che le aziende hanno posto in essere su questi grandi mercati, nei quali se in valore l'Italia non è ancora la prima

proprio quando quel prodotto in quei mercati comincia a essere conosciuto, la limitazione non gli consente di recuperare un vantaggio competitivo. Allora, ciò che chiedo al Governo è di cambiare impostazione e di eliminare

dia accesso ai programmi di promozione sui mercati terzi ponendo un limite temporale che non può essere fissato per legge. Dipenderà piuttosto dalla capacità con cui quell'azione riuscirà a determinare dei risultati.

ringrazio gli interroganti, la senatrice Ginetti e il senatore Gasparri, per la duplice opportunità fornita oggi al Dicastero, quella di delineare sinteticamente, ma con chiarezza i contenuti di un'iniziativa senz'altro importante in tema di sicurezza e quella di condividere in modo altrettanto chiaro la posizione italiana al riguardo, dissipando le apprensioni che questa scelta potrebbe aver provocato. La European intervention initiative - Iniziativa di intervento europeo, volendola definire in italiano è stata promossa dalla Francia con l'obiettivo di sviluppare, attraverso la condivisione di informazioni, una cultura strategica comune ai Paesi che vi aderiscono, al fine di facilitare, se necessario, la rapida attivazione di operazioni per la salvaguardia di interessi strategici condivisi in maniera svincolata dalle dinamiche decisionali dell'Unione europea e della NATO. Nello specifico, l'iniziativa mira a sviluppare legami tra le Forze armate di alcune Nazioni europee, selezionate in base ai criteri della disponibilità di capacità militare e della volontà politica di agire, coinvolgendole in settori chiave la *situational awareness* (analisi di scenari), il supporto operativo e lo sviluppo della dottrina e delle lezioni apprese. Il progetto, quindi, non promuove la costituzione di una forza, né tende a formare le cosiddette forze armate della UE, né comandi, né assetti per interventi militari. Questa iniziativa, dopo un periodo di negoziazione seguito dal precedente Governo, è stata ufficializzata con una lettera di intenti che i Ministri della difesa di Francia, Germania, Belgio, Regno Unito, Danimarca, Olanda, Estonia, Spagna e Portogallo hanno firmato lo scorso 25 giugno in Lussemburgo. Il progetto è ancora nella sua fase embrionale e molto è ancora da definire. Sussistono, tuttavia, sufficienti elementi per una sua valutazione di merito e di opportunità. Nel merito, pur condividendone la finalità principale, ossia il creare una comune cultura strategica europea, sarebbe tuttavia prematuro, considerati gli interessi in gioco, aderire all'iniziativa senza averne prima ponderato l'impatto su importanti progetti comuni già consolidati o in fase di avvio in ambito europeo nel settore della sicurezza e della difesa. In particolare, sul piano politico un'analisi dei contenuti della proposta fa emergere il concreto rischio che a essere tutelati siano i soli interessi strategici degli Stati aderenti all'iniziativa, interessi che, tuttavia, possono non coincidere con quelli dell'Unione europea nel suo complesso che proprio l'Italia, al contrario, sta cercando con fatica di far promuovere nella direzione di un'autonoma e concreta capacità di difesa da parte dell'Unione. Sussiste, in altri termini, il rischio di una frammentazione in un'Europa a due velocità: da una parte il gruppo degli Stati selezionati che aderiscono alla proposta; dall'altra quelli che ne restano fuori. Da tale frammentazione potrebbero risultare compromesse sia la credibilità della coesione dell'Unione europea in questo delicato settore sia l'impegno italiano, unanimemente percepito e riconosciuto, nella costruzione di un'unione politica con una forte competenza di sicurezza e difesa. Passando all'aspetto strettamente tecnico dell'iniziativa, si evidenziano ulteriori potenziali criticità che è necessario approfondire e che sono correlate al pericolo di una duplicazione e dispersione di risorse, nonché alla possibile sovrapposizione a strutture e a meccanismi similari già esistenti o di prevista prossima creazione non solo in ambito UE, ma anche in quello NATO e multinazionale, con potenziali sprechi di risorse da evitare. Sul piano dell'opportunità, l'ufficializzazione della European intervention initiative ci sembra non essere del tutto in sintonia con il particolare momento politico che sta vivendo la tanto agognata difesa europea, che vede finalmente

Onorevoli senatori, come credo risulti evidente da quanto ho detto, questo Governo non si oppone, in linea di principio, alle finalità perseguite dalla European intervention initiative, se orientate allo sviluppo di una cultura strategica integralmente europea e se a salvaguardia di interessi strategici realmente comuni. In questo senso siamo attenti a coglierne ora i concreti sviluppi, valutandone progressi e risultati per eventuali nostre decisioni future. Nello stesso tempo - e mi rivolgo a quanti, temendo l'isolamento nazionale, considerano *a priori* l'iniziativa come un treno da non perdere - non possiamo ignorare ciò che è emerso dal lungo lavoro dedicato al perfezionamento della lettera di intenti condotto dal precedente Governo. Mi riferisco al rischio di una possibile sovrapposizione con la PESCO, una realtà naturalmente inclusiva e orientata a perseguire i fini e gli interessi di tutta l'Unione europea. Per questi motivi l'Italia, ritenendo molto più remunerativo operare dall'interno dell'Unione per per il miglioramento degli strumenti disponibili, ribadisce, almeno per il momento, il proprio prioritario impegno nei progetti PESCO, nel cui ambito ritiene molto più utile includere l'iniziativa in parola.

Dal punto di vista del merito, non c'è alcuna contrapposizione con l'attività della neo-PESCO, quindi di una cooperazione strutturata permanente, anzi, al contrario, l'iniziativa europea l'iniziativa europea di intervento è strettamente collegata all'attività della PESCO ed è a supporto della stessa, tant'è che questi nove Paesi europei, a margine del Consiglio, il 25 giugno, hanno deciso di progredire nell'ipotesi di una cooperazione rafforzata

partecipare a questa presa di posizione, a questa evoluzione verso una comune difesa europea, nell'ambito, tra l'altro, di quanto previsto dallo stesso Trattato di Lisbona. Vorrei ricordare, in particolare, che significativi progetti di ricerca sono stati già assegnati appunto nei settori dell'industria e della ricerca in materia di difesa e che il più importante di questi quattro progetti è stato attribuito ad un consorzio guidato da una società italiana. Quindi, anche da questo punto di vista, è estremamente importante far parte di un contesto di programmazione di questa evoluzione, constatato che si dovrebbe poter contare su 500 milioni milioni di euro per il prossimo biennio 2019-2020. Pertanto, il nostro auspicio è che, proprio l'evoluzione rispetto

Questa parziale risposta poteva essere data dal Governo, in quanto questa nostra assenza ha creato disorientamento in una fase in cui non dobbiamo dimenticare quanto sia difficile la nostra presenza nell'ambito delle istituzioni europee, dove talvolta con ragione abbiamo rivendicato politiche diverse sul fronte della difesa e della sicurezza e anche dell'impiego di strutture della Difesa. Pensiamo al fronte sul meridionale d'Europa, quello del Mediterraneo, che poi con l'ingresso dei clandestini causa le tensioni intraeuropee sui famosi passaggi di secondo grado: se uno entra in Europa, cerca di passare dall'Italia all'Austria o dall'Austria alla Germania, ma se non ci fosse l'ingresso l'ingresso principale al confine d'Europa non avremmo il problema del transito secondario. A nostro avviso quindi tutte le iniziative che puntano a un maggiore raccordo

sindacato ispettivo noi abbiamo suscitato un primo parziale chiarimento, perché la risposta ci indica qualche elemento riguardante la politica del Ministero della difesa, che sin qui è stato un oggetto misterioso. se si esclude l'intervista rilasciata in data odierna dal Ministro della difesa sul giornale «Avvenire», non abbiamo ancora avuto le comunicazioni di avvio legislatura, anzi di avvio mandato; in questo caso il mandato del Governo e l'avvio di legislatura, un po' in ritardo per le note vicende, coincidono noi non sappiamo ancora quale sarà l'indirizzo. Oggi c'è un'intervista che riguarda alcune questioni, come la sentenza della Corte sul sindacato che si dovrà istituire e il tema dell'uranio, con tutte le conseguenze sul personale della Difesa; noi vorremmo però capire quali sono gli orientamenti generali. Abbiamo in discussione acquisti e e investimenti che riguardano i droni con possibili ricadute negative, in base alle decisioni che verranno prese, su impianti industriali italiani, su rapporti internazionali, su prassi di difesa e di sicurezza.

di difesa, una questione che da decenni l'Europa discute e che può essere anche portatrice di una razionalizzazione delle spese, di interventi che possano liberare risorse per il personale o per diverse esigenze di sicurezza. Insomma, noi vorremmo sapere anche su questo aspetto quale sia la politica del Governo; finora c'è stata la non partecipazione, dopo un interesse manifestato dall'Italia in un'altra fase, a questa iniziativa a nove tutti i principali Paesi europei, ma l'Italia non c'è stata; anche se è qualcosa in fieri, anche se è qualcosa che deve avere una sua definizione nel futuro, è bene esserci per annusare l'aria, per capire dove si va e indirizzare i processi. Noi sollecitiamo quindi il Governo ad una maggiore presenza in queste iniziative; poi la storia ci dirà quali saranno quelle che avranno sviluppo, se i progetti di difesa europea avranno uno sviluppo reale o se saranno tentativi destinati ad avere poco successo. Di questo tema, del resto, si discute fin dai tempi del generale De Gaulle con molti fallimenti e scarsissimi successi. Concludo, signor Presidente, augurandomi che le

ma anche la Marina e la Guardia costiera che portano clandestini. Non sono un profeta, ma, seguendo queste vicende, avevo detto quello che si sa verificando in queste ore. La politica della difesa è connessa anche a quella di sicurezza e di contrasto all'immigrazione. Vorremmo capire se tutti i Ministri hanno le stesse idee e la stessa politica.

per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno il senatore Berutti pone l'attenzione sulla situazione del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Alessandria e chiede se il Governo sia a conoscenza della carenza di personale che interessa quel comando e quali iniziative si intendano adottare, anche in relazione alla complessiva dotazione organica del Corpo nazionale nella regione Piemonte. In via preliminare, mi preme sottolineare che questo Governo riserverà una particolare attenzione alle problematiche concernenti il potenziamento di uomini e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, al momento, a fronte di una previsione organica di 37.481 dipendenti, soffre una carenza di poco più di 3.000 unità. Al riguardo, sono in corso di attuazione alcune misure volte a mitigare l'incidenza di tale *deficit*. Mi riferisco, in particolare: all'autorizzazione a bandire una nuova procedura selettiva per l'immissione di 250 giovani nella qualifica di vigile del fuoco; all'assunzione straordinaria di 1.300 unità, con una programmazione quinquennale, a decorrere dal 1° ottobre di ogni anno: per il 2018 sono previste 50 assunzioni; all'assunzione di 400 unità nei ruoli iniziali del Corpo nazionale, già avvenuta in data 7 maggio scorso, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al cento per cento delle cessazioni avvenute nel 2017: gli allievi vigili hanno già iniziato l'ottantatreesimo corso di formazione che avrà termine entro la fine dell'anno; ad un incremento della dotazione organica della qualifica di Vigile del fuoco di 300 unità con decorrenza 1° ottobre 2018. Occorre, inoltre, evidenziare che il Corpo è stato chiamato a fronteggiare maggiori oneri funzionali in virtù di recenti interventi normativi come, ad esempio, la lotta attiva agli incendi boschivi dopo l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato o l'assunzione di un ruolo di coordinamento tecnico-ispettivo negli interventi di soccorso pubblico più complessi, sancito anche nel nuovo codice della Protezione civile, nonché i più onerosi impegni che scaturiscono dalle nuove direttive sulla sicurezza integrata in occasione delle manifestazioni pubbliche. Tali circostanze determinano, effettivamente, la necessità di prevedere l'immissione di ulteriori unità di personale per assolvere adeguatamente anche alle nuove missioni prima delineate. Segnalo, inoltre, che è stato recentemente licenziato dal Consiglio dei ministri, in via preliminare, un intervento normativo che porta a compimento il disegno riformatore iniziato nel 2017 e che mira a garantire l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale nonché l'implementazione dell'assetto ordinamentale del relativo personale. È un intervento molto complesso che si rivolge all'intera compagine operativa, attraverso la valorizzazione di tutte le risorse umane e delle loro professionalità. L'intervento complessivo, peraltro, comporterà una revisione del dispositivo territoriale con l'istituzione dei distretti - unità organizzative intermedie tra comandi e distaccamenti - soprattutto nelle realtà industriali o più fortemente antropizzate su base distrettuale, suscettibile di rendere più efficace la risposta operativa del Corpo nazionale. Si tratta di un'innovazione che avrà conseguenze positive su tutti i territori di riferimento in quanto assicurerà, anche per gli aspetti di prevenzione, una maggiore vicinanza dell'amministrazione alle esigenze della cittadinanza e delle imprese nelle materie di competenza istituzionale. Venendo, in maniera più specifica, all'atto dell'interrogazione, rappresento che il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Alessandria, a fronte di una dotazione organica teorica pari a 292 unità (di cui 4 direttivi, 2 sostituti direttori, 8 ispettori antincendio, 20 capi reparto, 70 capi squadra, 164 vigili del fuoco e 24 unità amministrativo-contabili e tecnico-informatiche), presenta un organico di 249 unità (di cui 3 direttivi, 4 ispettori antincendio, 20 capi reparto, 53 capi squadra, 153 vigili del fuoco e 16 unità di personale del ruolo amministrativo e tecnico informatico). Con particolare riferimento al personale operativo, si evince che, mentre per la qualifica dei capi reparto si registra la piena copertura dell'organico, per i capi squadra la carenza è pari al 24 per cento, superiore alla media nazionale che è del 13,65 Per il ruolo dei vigili la carenza è, invece, del 6,7 per cento, rispetto alla dotazione nel medesimo ruolo che, a livello nazionale, presenta una lieve carenza, pari allo 0,3 Complessivamente, la carenza di tutto il personale operante presso il comando di Alessandria, è pari al 14,72 per cento, superiore a quella nazionale, pari al 7,28 per cento. Tenuto conto di tale situazione organica, nel maggio scorso, a seguito della conclusione dell'81° corso

prossimo venturo, sarà prevista l'assegnazione agli uffici territoriali, dei vigili provenienti dall'82° corso di formazione, mentre nel mese di settembre saranno avviate le procedure per la ricognizione e la successiva assegnazione dei vigili provenienti dai corsi 83° e 84°. Inoltre, per quanto attiene al ruolo dei capi squadra e capi reparto, si rappresenta che è in via di definizione la procedura di promozione alla qualifica di capo squadra che riguarda 608 unità. In relazione a quanto, poi, richiesto dall'interrogante circa la dotazione organica relativa alla regione Piemonte, evidenzio che per quanto concerne il personale operativo, a fronte di una dotazione teorica di 1.901 1.901 unità si registra una presenza effettiva pari a 1.717 unità con una carenza del 9,68 per cento superiore a quella nazionale che è pari, complessivamente, al 3,53 Faccio presente, infine, che il soccorso sul territorio provinciale è comunque garantito con professionalità ed efficienza, anche modulando l'organizzazione con l'intervento, ove necessario, delle squadre provenienti dai territori più vicini. A conclusione, aggiungo anche che sarà, come già accennato, impegno e onere del Governo presentare al Parlamento un piano assunzionale che vada ulteriormente a ridurre le difficoltà di organico, badando ovviamente a che il Parlamento abbia intenzione di approvare tali richieste di provvedimento.

in questi anni, in quest'ultimo periodo, nella rivoluzione portata avanti in merito al Corpo forestale, al cambiamento, anche climatico, ormai epocale e a tutta una serie di situazioni contingenti, è chiara la necessità di fare un lavoro strutturale. E diciamo che io apprezzo anche la visione più ampia. Io mi sono soffermato sostanzialmente sulla regione Piemonte, su un problema legato alla mia provincia ma,

Mi sembra che siamo, in questa fase, in una situazione abbastanza debole in termini di proiezione e in termini di assunzioni. Mi rendo poi conto che siamo in una fase iniziale e, pertanto, l'auspicio è quello che, in base al programma che verrà posto si parli di numeri

ventinovenne Duccio Dini travolto, lo scorso 10 giugno 2018, a Firenze, nella zona di via Canova, mentre si trovava sul proprio *scooter* fermo al semaforo, semaforo, da un'auto impegnata in un inseguimento scaturito dopo una violenta lite per contrasti nei rapporti familiari tra soggetti di etnia rom, alcuni dei quali residenti nel campo del Poderaccio. Sull'episodio, che ha suscitato grande commozione, si sono concentrate fin dall'immediatezza dei tragici eventi le indagini del comando provinciale dei Carabinieri di Firenze, che hanno portato all'identificazione di quattro persone risultate coinvolte nel fatto, fatto, già conosciute alle Forze di polizia per aver commesso infrazioni penali o essere state sottoposte a controlli di polizia sul territorio. Tra queste, due persone sono state arrestate per il reato di lesioni personali gravissime in concorso, rubricato poi dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze in omicidio doloso in concorso, reato per il quale si trovano tuttora detenuti presso la casa circondariale di Firenze-Sollicciano. Una terza persona è stata denunciata a piede libero per il reato di lesioni personali gravissime in concorso, anch'esso rubricato poi in omicidio doloso in concorso e, successivamente arrestata, il 4 luglio scorso. Nella medesima data, i carabinieri del comando provinciale di Firenze hanno arrestato altre tre persone in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip presso il tribunale di Firenze su richiesta della locale procura della Repubblica, nei confronti di soggetti di etnia rom. Come accennato in precedenza, le due persone arrestate nell'imminenza del fatto risiedono nel campo rom del Poderaccio - più precisamente denominato Villaggio rom del Poderaccio I e II lotto - dove, attualmente, vivono 242 persone di cui 79 minori, delle quali, come riferito dal comando provinciale dei Carabinieri, 76 sono gravate da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona, in materia di stupefacenti e altro. L'amministrazione comunale di Firenze ha, altresì, informato che le presenze all'interno del campo, in questi ultimi anni, sono state dimezzate e che uno degli obiettivi del Comune è la chiusura definitiva del Poderaccio, prevista in un arco temporale di diciotto Nel corso degli ultimi mesi sono state già operate azioni di allontanamento di persone non autorizzate, di abbattimento di alcuni manufatti edificati abusivamente e di controllo anche sulla regolarità dei veicoli presenti. In merito ad altre due persone arrestate in un secondo momento, lo stesso Comune di Firenze ha rappresentato che esse risiedono in altrettanti alloggi popolari, posti in via Simone Martini e in via Attavante, e che per le medesime non risultano segnalazioni o denunce per episodi di violenza o di disturbo. Per quanto concerne le modalità di assegnazione delle unità di edilizia residenziale, lo stesso ente comunale ha precisato di non disporre di classificazioni per etnia degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di attribuire le case popolari secondo, i criteri dettati dalla disciplina vigente. In caso di denunce che attestino episodi di violenza all'interno del condominio o gravi violazioni delle norme condominiali, l'amministrazione comunale procede con le decadenze, come consentito dalla normativa di riferimento. La legge regionale sull'edilizia residenziale pubblica (n. 96 del 1996), infatti, permette di dichiarare la decadenza dell'assegnazione quando l'assegnatario «abbia gravemente e reiteratamente contravvenuto alle disposizioni di legge, di regolamento di utenza e del regolamento di autogestione inerenti l'uso dell'alloggio, o abbia causato volontariamente gravi danni all'alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni dell'edificio». L'ordinata convivenza negli edifici di edilizia residenziale pubblica è assicurata, secondo il Comune, dal continuo sviluppo del sistema delle autogestioni, che vengono incoraggiate e sostenute dall'amministrazione comunale in tutte le situazioni ove ciò è possibile, anche attraverso il monitoraggio da parte dell'amministrazione medesima. Informo che sono in corso di revisione, da parte del Comune, le posizioni di alcune famiglie prima residenti nel campo citato, che hanno potuto accedere agli edifici di edilizia residenziale pubblica. Riguardo, poi, alla richiesta di chiarimenti avanzata dall'interrogante circa la mancata applicazione, nei confronti dei soggetti coinvolti nella vicenda, del cosiddetto Daspo urbano, va evidenziato che il Comune di Firenze ha rilevato che la citata misura di allontanamento può essere disposta, in base alla normativa vigente, solo per specifiche aree, per alcuni definiti comportamenti e per un limitato arco temporale. Più in generale, sul fronte delle iniziative in tema di sicurezza e di controllo del territorio, informo che, dopo i fatti accaduti in via Canova, nella stessa serata del 10 giugno presso la prefettura di Firenze si è tenuta una riunione di coordinamento delle Forze di polizia, nell'ambito della quale è stata disposta l'intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo nei pressi dell'insediamento del Poderaccio. La questione è stata ulteriormente affrontata nella seduta del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 13 giugno ultimo scorso, alla presenza del sindaco di Firenze. Nell'occasione, il primo cittadino ha confermato che l'amministrazione ha già avviato il progressivo smantellamento di tale insediamento e che, nelle more del suo completo svuotamento, attiverà un'azione di controllo H24. Infine, sul tema della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica sul territorio dell'area metropolitana fiorentina, assicuro che la situazione è costantemente monitorata dalla competente prefettura, attraverso sedute settimanali del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e riunioni di coordinamento delle Forze di polizia, dove vengono esaminate tutte le problematiche emergenti. In particolare, le Forze di polizia sono attente ad intercettare ogni minimo segnale di rischio per la sicurezza dei cittadini e, per soddisfarne la legittima domanda, i servizi di prevenzione generale, nel corso di apposite riunioni tecniche interforze e in base alle criticità riscontrate, vengono di volta in volta rimodulati e intensificati attraverso mirati piani di controllo. Concludo, signor

Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli senatori, prendiamo atto della sua risposta, che non poteva ovviamente entrare nel merito di alcune questioni poste nell'interrogazione, perché si fa riferimento ad alcune enunciazioni di principio da parte del Comune di Firenze. quello che è avvenuto per quanto riguarda la morte di Duccio Dini ha dell'incredibile, perché è la punta dell'*iceberg*, è la fase finale di un'*escalation* che si è verificata nella città di Firenze (ma si poteva verificare in qualsiasi altra parte del nostro territorio nazionale) e in cui c'è qualcuno che, nelle nostre città, pensa di essere al di sopra della legge, di non rispettare le regole e di fare quello che gli pare. E, quando inizia questo percorso, in cui qualcuno si sente al di sopra della legge e nella possibilità di fare quello che gli pare quindi di non rispettare le regole della civile convivenza, poi si arriva anche al punto finale, in cui: che male c'è se si fa un inseguimento? Non era la prima volta che veniva svolto un inseguimento per le strade cittadine, in cui, in una sorta di *far west*, ci si insegue per fare un regolamento di conti; poi ci lascia la pelle un povero ragazzo che quel giorno stava andando a lavorare. Questa è la fase finale di una situazione di illegalità che continua nel tempo, che non ha freno. La cosa più grave, che pongo alla vostra attenzione, signori del Governo, è che abbiamo visto dare a questi signori anche le case popolari, come anche lei ha rilevato nel suo intervento. Nel Comune di Firenze non c'è solo il problema del campo nomadi del Poderaccio,

ladro, facevano vedere biglietti da 50 euro essendo degli usurai, perché hanno precedenti penali vari, e il Comune di Firenze gli ha dato le case popolari. È incredibile! Di fronte al fatto che ci sono tantissime famiglie nella mia città, Firenze, che chiedono la casa popolare, che non hanno

che dovete intervenire, al di là delle enunciazioni di principio che state facendo in questi giorni, su fatti concreti. Nella scorsa legislatura il centrosinistra ha approvato le cosiddette leggi svuotacarceri. Gli ultimi provvedimenti e decreti attuativi sono stati fatti dal Governo Gentiloni Silveri addirittura durante la campagna elettorale e prevedevano l'impunità per moltissimi reati che vengono imputati a questi soggetti, per cui truffare, derubare e entrare in casa delle persone ormai non sono più reati che si scontano con il carcere e la pena detentiva, ma con con gli arresti domiciliari o l'affidamento in prova e in Toscana abbiamo avuto situazioni di persone fermate e portate davanti al giudice per 200, 300 volte e rimandate agli arresti domiciliari. Il giorno dopo escono e vanno a fare i furti. Basta!

con il giovane Duccio Dini, che ha perso la vita quel giorno, mentre andava a lavorare. Tutti a Firenze lo piangono, i cittadini e i suoi familiari, e secondo me è una disgrazia che si poteva evitare.

l'effetto provocato dalla sentenza del Consiglio di Stato del 15 giugno 2018, n. 1546. Stiamo parlando del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente ulteriori modifiche al decreto

che in origine concernevano esclusivamente chi aveva compiuto diciotto anni nel 2016 e nel 2017. Dopo il parere del Consiglio di Stato, una parte dei contenuti già propri della legge di stabilità trova ora collocazione nella II sezione della legge di bilancio, in particolare per quanto riguarda la possibilità di disporre il rifinanziamento,

Proprio per sopperire alla predetta mancanza normativa e consentire l'utilizzo dei fondi che sono già stati accantonati e sono in legge di bilancio, la proroga del *bonus* cultura per gli anni 2018 e 2019 verrà disciplinata mediante apposito decreto-legge, che a breve invieremo al Consiglio dei ministri. alcuni numeri per chiarire di cosa stiamo parlando. Nel primo anno di vita, il 2016, il Ministero ha trasferito alla Consap 165 milioni di euro a fronte di una copertura finanziaria che per ogni anno è di 290 milioni di euro, il che vuol dire che in un anno non abbiamo utilizzato 125 milioni di euro e, personalmente, penso che questa sia una grave mancanza di utilizzo di risorse pubbliche. Per il 2017 sono già stati trasferiti 100 milioni di euro - ma il dato è ancora parziale - e, nonostante questo, mi aspetto che gran parte delle somme accantonate non sarà spesa.

Senza *vis* polemica, vorrei ricordare che la possibilità di acquistare libri non era prevista originariamente nel disegno di legge, ma è stata permessa da un emendamento del MoVimento 5 Stelle,

Rimangono le perplessità riguardo al *bonus* cultura. Ricordo che tale *bonus* non ha nulla di strutturale, ma viene deciso anno per anno; non prevede misure premiali e non tiene conto delle diverse situazioni delle famiglie. Per questo motivo è intendimento di questo Ministero predisporre un programma strutturale per la promozione del consumo culturale, che associ progetti di diffusione della cultura nelle scuole con incentivi agli acquisti di prodotti e servizi, a partire dal 2020. Il *bonus* cultura verrà rimodulato e corretto in modo da pianificare misure a lungo termine tali da stimolare la ricerca di cultura fra i giovani, non solo diciottenni, ed evitare le distorsioni verificatesi nel passato. Alla predisposizione delle necessarie modifiche provvederà un'apposita commissione di esperti che, partendo dall'analisi di come i fondi sono stati utilizzati e dopo aver recepito le esigenze di tutte le persone e i soggetti coinvolti, individuerà i correttivi indispensabili per assicurare al *bonus* cultura un ruolo fondamentale nello sviluppo della cultura tra i giovani.

non sono per nulla soddisfatta, perché c'è un'impostazione culturale che lei continua a ribadire, al netto del fatto che questa interrogazione è stata fatta anche a fronte di una serie di sue affermazioni che ci avevano lasciati

ai nostri ragazzi, mentre noi pensiamo che uno Stato - è una visione culturale, è un'impostazione - debba invece spingere al consumo dei beni culturali e all'accesso alla cultura. Parlavo

perché non è la prima volta che nei suoi interventi, come ha fatto anche garbatamente ieri in audizione esponendo le sue linee programmatiche, ribadisce che è necessario considerare anche la situazione delle famiglie. Non è detto che provenire da una famiglia benestante sia necessariamente chiave per far accedere un ragazzo alla cultura. Noi riteniamo che sia importante un'impostazione che garantisca che lo Stato dia questo diritto di cittadinanza culturale ai nostri ragazzi.

le auguro di poter lavorare nella modalità più serena possibile però, quando lei vorrà applicare una misura così importante quale il *bonus* cultura o qualsiasi altra misura che uscirà dal suo Ministero, si ricordi che tra il poterla realizzare e la fase di realizzazione c'è un abisso. Noi abbiamo provato in via sperimentale a dare un segnale che andasse in quella direzione, tenendo ben conto dei risultati e apportando alcune modifiche

per due ragioni. La principale ragione è che lei ha dichiarato chiaramente in quest'Aula la prossimità di un decreto-legge per confermare intanto quanto oggi presente in legge di bilancio.

possono sempre avere il tempo che trovano, ma soprattutto in discontinuità con la posizione delle forze che appoggiano questo Governo nella scorsa legislatura, che erano pesantemente contrarie a questo provvedimento.

siamo disposti e intenzionati a cambiare posizione su alcuni aspetti. Se qualcuno mi facesse la domanda: si può migliorare il *bonus* 18app? Direi: assolutamente sì. Lei ha fatto un'osservazione puntuale sulle risorse che

Siamo riusciti a prorogarlo per tre anni. Se oggi stiamo discutendo di questo è perché siamo riusciti a trovare questi fondi e naturalmente saremo, come ha detto la collega Malpezzi, assolutamente dalla sua, se ci sarà possibilità in legge di bilancio di stabilizzarlo per sempre, anche perché ormai considereremmo un'ingiustizia che tre generazioni di italiani, casualmente nate in un determinato anno, abbiano potuto usufruire di questo e quelle successive, misteriosamente, no. Pertanto, conduciamola insieme, questa battaglia. un altro punto. Sicuramente il tema della scuola è importante, però stiamo attenti a non confondere i due aspetti. Noi le abbiamo lasciato in eredità un bene prezioso e lo abbiamo lasciato in eredità anche con il voto favorevole o con un'astensione benevola di chi allora era in minoranza: i decreti attuativi della legge sullo spettacolo dal vivo. Tra quei decreti attuativi e in quella legge ci sono risorse dedicate per portare le attività culturali e lo spettacolo dal vivo nella scuola. È una cosa fondamentale. I decreti scadono e c'è una preoccupazione per questa scadenza. Lei ieri si è preso l'impegno di riuscire, entro il mese di dicembre, ad attuarli; le daremo una mano, se è possibile. Le daremo anche una mano se sarà necessaria una proroga breve, perché ci rendiamo conto non siamo qui a scherzare. È una grande opportunità per il Paese, ma 18app o qualsiasi misura che lavora sul fronte della domanda culturale è qualcosa di diverso rispetto a ciò che si può fare a scuola. Glielo dico con il cuore, glielo dico così: spesso quello che ci insegnano a scuola lo viviamo in maniera pregiudiziale, come qualcosa che, che, venendo dall'autorità e dalle istituzioni, non ci piace. Quando siamo ragazzi, siamo un po' così, siamo un po' ribelli, vogliamo scegliere noi e 18app è la possibilità per i ragazzi di scegliere loro, liberamente, senza essere giudicati. Hanno scelto moltissimi

riflettiamo veramente, guardiamoci negli occhi, facciamolo da persone prima che da politici di parte. Io ero dell'opinione che dovessimo differenziare questo intervento sulla base del reddito delle famiglie di provenienza; ho cambiato idea, ho cambiato idea, perché sono convinto che non è detto che un ragazzo proveniente da una famiglia benestante abbia l'appoggio dei genitori benestanti per i suoi consumi culturali, che magari vanno in direzione ostinata e contraria rispetto a quelle che sono le convinzioni dei suoi genitori. non fare differenza su ragazzi di diciotto anni, perché i ragazzi di diciotto anni non sono né benestanti, né in condizioni di povertà: non sono ancora in nessuna di queste due condizioni e questa è una grande opportunità. Chiudo, perché ho finito il tempo, dicendo: dedichiamo un tempo breve, ma intenso, per approfondire questa misura e facciamola diventare davvero un punto su cui questo Parlamento fa un salto di qualità, superando i pregiudizi di parte e i tanti luoghi comuni che

perché vi garantisco che in otto legislature non mi era mai capitato di assistere ad una seduta di interrogazioni con una partecipazione che equivale veramente a quella totale di un trentennio. È stata anche una seduta svolta in maniera corretta ed educata: chissà che questo cambiamento non parta dall'istituzione Senato.